è senz'altro costituito dall'intervento del ministro della giustizia Alfano al convegno Ambrosetti di Cernobbio dei primi di settembre. In quell'occasione il ministro Alfano, davanti a una platea qualificatissima e alla stampa internazionale, ha dichiarato che non intendeva reintrodurre la regola dei minimi inderogabili nelle tariffe relative alle libere professioni. Ha detto ciò non in riferimento a una sollecitazione generica, ma di fronte a una domanda che gli veniva rivolta dall'avvocato Maurizio de Tilla, presidente dell'Organismo unitario dell'avvocatura. non c'è dubbio che il Ministro abbia inteso riferirsi anche alla riforma che è all'esame del Senato in questo momento. non vi è niente di disdicevole nel fatto che il Governo possa esprimere un parere negativo su una parte di un disegno di legge di iniziativa parlamentare che in questo caso - e ovviamente solo in questo - il Governo avrà il nostro pieno appoggio. Su questo punto occorre però fare chiarezza quindi chiedo che il Governo dica chiaramente, in questa sede e adesso (non in un altro momento), quali sono i suoi intendimenti riguardo a questa disposizione, che ha un valore cruciale e direi in qualche modo emblematico in riferimento all'intera riforma. Forse disdicevole sarebbe semmai che il Governo tacesse su questo punto, come ha fatto stamattina di fronte a una mia prima sollecitazione. Ripeto: occorre chiarezza. Se il ministro Alfano a Cernobbio ha detto una cosa e adesso ne pensa un'altra, che lo dica: anche in questo non ci sarebbe niente di male. Quello che non è ammissibile è che su un punto di questa importanza ci sia un grave difetto di chiarezza, un atteggiamento furbesco e doppio. Detto questo, io credo che avesse pienamente ragione il ministro Alfano nel prendere quella posizione. In realtà non è affatto vero

Non è vero che la regola dell'inderogabilità dei minimi avvantaggia soltanto le grandi imprese o le banche. Intendiamoci, se anche fosse vero che se ne avvantaggiano le grandi imprese, in questo non vedrei niente di male, dal momento che è noto che in Italia le imprese sono penalizzate rispetto alle loro concorrenti internazionali per un più alto costo dei servizi - e tra questi c'è anche il servizio legale rispetto a quanto accade negli altri Paesi e questo accade proprio per un difetto di concorrenza nel corrispondente mercato italiano. non ci sarebbe proprio motivo di rammaricarsi se quella piccola rendita generata dalla limitazione della concorrenza venisse abolita a vantaggio delle imprese. Il punto però è che in realtà a soffrirne è anche l'uomo della strada, è anche la povera gente. A questo proposito, vorrei raccontarvi molto brevemente una mia esperienza personale vissuta di responsabile del coordinamento dei servizi legali della Camera del lavoro di Milano, in un'epoca in cui la regola dell'inderogabilità dei minimi era La Camera del lavoro di Milano stabilì in modo molto esplicito un sistema di remunerazione dei propri legali, di quelli cioè che operavano in collegamento stessa Camera del lavoro, in cui sostanzialmente si prevedeva un acconto molto ridotto, eravamo negli anni '70 si chiedevano 20.000 lire per l'inizio della pratica, e poi si chiedeva al lavoratore di destinare a remunerare l'avvocato il 5 per cento di quanto eventualmente recuperato con la la vittoria in giudizio se il giudice non avesse provveduto a condannare la controparte alle spese: era quello che si chiama il patto di quota lite.

Pubblicammo apertamente questa regolamentazione e poco dopo venni convocato dal presidente del consiglio dell'ordine, che era allora Giuseppe Prisco, il quale mi disse: «Caro Ichino, non si può fare, la disciplina della materia lo vieta»; io gli risposi: «Benissimo, metteteci tutti sotto procedimento disciplinare, voglio farne una battaglia fino ad arrivare davanti alla Corte costituzionale, perché o facciamo in questo modo oppure i servizi legali agli operai non si possono offrire in termini realmente accessibili».

decisero di lasciar correre, con la raccomandazione di non dire troppo in giro che le cose funzionavano in quel modo. Noi non accogliemmo neanche quella raccomandazione, continuammo a farlo alla luce del sole; però era una violazione evidente della vecchia regola sull'inderogabilità Allora cosa vogliamo fare? Vogliamo davvero tornare al principio del «si fa ma non si dice»? Vogliamo davvero tornare ad un regime in cui il lavoratore che deve recuperare 100 o 1.000 euro deve sborsare per la causa un minimo che comunque rende impraticabile l'azione legale? Di questo si tratta nella questione ci sta anche la regola sul divieto di patto di quota lite, la quale per quel tipo di cause è sostanzialmente inevitabile. lo è ancora di più nel momento in cui si introduce davvero nel nostro sistema la *class action*. Tutti sanno che quest'ultima non può funzionare se non raccogliendo adesioni in gran numero all'iniziativa giudiziaria sulla base di un patto di quota lite. Allora come la mettiamo: vogliamo la *class action* da una parte, ma rifiutiamo la condizione indispensabile

che vive difendendo vecchie, piccole o grandi rendite e poi, invece, legare le mani dietro la schiena alla parte più dinamica

per competere ad armi pari e quindi di raccogliere i capitali necessari attraverso la società per azioni. Si sta facendo un'operazione regressiva, che non va nell'interesse dell'avvocatura e ancor meno va nell'interesse del Paese.

Presidente, mi preme soltanto illustrare l'emendamento 12.225, che vorrei modificare in parte perché,

che attribuiscono all'avvocato una quota del risultato della controversia sono consentiti nei casi in cui si esercita l'azione di classe ai sensi dell'articolo 140-*bis* del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206».

collegarmi al discorso del senatore Ichino. La *class action*, senza che si preveda la possibilità che all'avvocato sia attribuita una quota del risultato della controversia, non può essere esperita in questo Paese,

opportuna, attuale, anzi necessaria la proposta che una quota del risultato della controversia sia attribuita all'avvocato che esercita l'azione di classe. di classe. Nello stesso concetto di azione di classe è insita sostanzialmente la previsione di base che l'avvocato possa essere cointeressato, naturalmente senza che ciò

una complessa serie di audizioni e di confronti. Sono del parere che il nostro sistema, come venga individuato in questo disegno di legge, debba continuare a prevedere

su proposta del Consiglio nazionale forense, sentiti il CIPE e il Consiglio di Stato. Il fatto che il sistema tariffario venga determinato con decreto ministeriale consente di superare il motivo principale delle critiche che sono state mosse in Europa al sistema italiano. Infatti, l'accusa che veniva fatta al nostro Paese, spesso con superficialità, era quella di ritenere il sistema tariffario frutto di una determinazione corporativa, a discapito quindi della concorrenza e senza il controllo di altre autorità.

la disciplina che andiamo ad approvare in contrasto con le norme sulla concorrenza e sul diritto di stabilimento.

le parole «tranne che nelle particolari ipotesi disciplinate dalle tariffe». In questo modo, nel momento in cui le tariffe sono determinate dal decreto ministeriale, sentite le autorità menzionate al comma 1 dell'articolo 12, si sfugge alla critica che può farci l'Europa per avere noi introdotto in una legge dell'ordinamento professionale un criterio rigido di applicazione delle tariffe. di vista le tariffe minime e massime sono inderogabili a pena di nullità, ma se il sistema tariffario dovesse prevedere delle ipotesi eccezionali, la la deroga è possibile, ovviamente in quelle ipotesi espressamente previste dal sistema tariffario approvato con decreto ministeriale. In questo modo siamo sicuri di essere in linea con le decisioni approvate in Europa e con le procedure che l'Europa nel passato ha avviato Paese per violazione del diritto di stabilimento e quindi per violazione della concorrenza, aspetto che deve riguardare anche gli avvocati della Comunità europea. Questo è l'unico sistema - e lo segnalavo quindi alla maggioranza e ai relatori - per cui la previsione di inderogabilità dei minimi e dei massimi diventa un criterio rigido, ma ritoccabile con rinvio alle ipotesi che dovessero essere previste dal regime tariffario introdotto con decreto

prevede tali possibilità di deroga ai minimi e massimi tariffari con rinvio proprio al regime tariffario

Intanto, vi è da ricordare - e questo se vogliamo è il paradigma all'interno del quale va inserito il ragionamento che quest'Aula è chiamata a fare - che l'obbligazione del professionista è obbligazione di mezzi e non di risultato,

che costantemente, anche dalla sua parte politica, viene invocato, non vedo di cosa potrebbe dolersi nel momento stesso in cui la sua domanda, giudicata dalla magistratura infondata, venisse respinta per i relativi costi della procedura. l'esempio da lei fatto relativamente all'esperienza della camera del lavoro di Milano mi pare inconferente. L'altro aspetto che vorrei segnalare, perché mi pare un po' contraddittorio, è il seguente.

tutte le componenti dell'avvocatura si sono riconosciute in un testo che già significativamente stiamo modificando e abbiamo modificato in Commissione, ha citato proprio quegli esempi che vanno nella direzione esattamente opposta rispetto a quella indicata

i colleghi, giovani o anziani, con la scatolina di cartone li mettono alla porta dalla sera alla mattina. Mi sembra dunque contraddittorio. Non c'è garanzia di sorta, e glielo dico per esperienze professionali anche dirette. Credo che anche da questo punto di vista

ponendo come proposizione iniziale l'espressione: «tranne che nelle particolari ipotesi disciplinate dalle tariffe».

semplificazione delle tariffe professionali, là dove si elimina la bipartizione di riti onorari e si va nel senso della semplificazione, auspicata anche dal CNF.

una breve dichiarazione di voto. Noi voteremo contro questo emendamento, in particolare con riferimento all'enunciazione contenuta nel riformulato comma 1. In realtà il comma 1*-bis* poi riporta il contenuto di quello riformulato include un divieto radicale di apposizione di condizioni rispetto al contratto al contratto che ha per oggetto l'incarico professionale. È ben vero che, di regola, il tipo di rapporto che sorge all'esito di questo tipo di contrattazione, per sua natura, non tollera o, in generale, non implica la posizione di condizioni. Il costringere, però, la mutevole complessità dell'esperienza giuridica e delle relazioni che possono intercorrere, di volta in volta, tra il cliente e l'avvocato con riferimento a vicende in cui l'incarico possa avere una natura preliminare e possa essere condizionato, nella sua estensione, al mutare della condizione giuridica, della controversia e dell'esigenza del soggetto interessato) denuncia una

vorrei approfittare di questa dichiarazione di voto per sollevare un problema che riguarda la qualità del confronto tra maggioranza, opposizione e Governo che stiamo sviluppando a proposito di questo disegno di legge. Signor Presidente, il professor Ichino poco fa nel suo intervento ha sollevato un problema preciso rivolgendosi al Governo. Ha citato una circostanza precisa: il recente convegno di Cernobbio, nel quale, non non qualcuno che passava lì per caso, ma il Ministro competente, cioè il Ministro della giustizia, ha sostenuto, di fronte a un uditorio qualificato e di livello internazionale, in presenza di un dibattito sopra la reintroduzione o meno delle tariffe minime, una posizione molto precisa di cui tutti gli organi di informazione italiana hanno dato notizia. Il Ministro ha detto: mi opporrò alla reintroduzione della norma relativa alle tariffe minime. Non voglio adesso Non voglio adesso discutere sopra il fondamento positivo o negativo, a mio giudizio, di questa posizione. Voglio sottolineare che, per la qualità del confronto pubblico, la presa di posizione del Ministro della giustizia su un tema tanto rilevante ha naturalmente un notevole peso. Questa posizione è stata richiamata dal senatore Ichino nel corso del nostro dibattito al fine di ottenere un chiarimento da parte del Governo, qui rappresentato autorevolmente dal sottosegretario

intendono essere favorevoli alla reintroduzione delle tariffe minime: è legittimo, ma va reso trasparente.

Una terza possibile posizione è la seguente: il Governo difende la posizione del Ministro, si rivolge alla sua maggioranza per ottenere un mutamento di parere del relatore di maggioranza. In ogni caso, signor Presidente, per la qualità del nostro confronto in questa sede, non può certo accadere che un senatore della Repubblica sollevi un problema, citando puntualmente una posizione presa dal Ministro, Ministro, ed il rappresentante del Governo di quello stesso Ministero finga di non avere ascoltato, perché questo rende del tutto inutile il confronto che stiamo facendo. Si rischia infatti che poi accada quello di cui tutti lamentiamo l'effetto e cioè che in questa sede non si dice nulla, poi magari si scopre che il Ministro

l'intervento del senatore Morando, in effetti, è stato svolto su un altro emendamento che riguardava altra materia. Invece l'emendamento in questione

Presidente. Francamente non sto rispondendo su sollecitazione del senatore Morando, perché è da un po' che chiedo la parola per rispondere a quello che mi aveva chiesto il senatore Ichino. Non intendo sottrarmi ad alcuna responsabilità. Non ero a Cernobbio e non so che cosa sia stato detto dal Ministro ma, dopo la discussione generale, dove ognuno ha esposto le posizioni in ordine a questo provvedimento, nel rispondere il Governo ha aderito *in toto* a questo impianto.

condivido il testo che ripristina sia i minimi tariffari, sia il divieto del patto di quota lite. Lo dico perché abbiamo sempre sostenuto che queste sono da un lato misure a salvaguardia della dignità professionale e dall'altro misure di trasparenza a vantaggio del cittadino utente. Tutti sanno che dove - ad esempio in America - il patto di quota lite è stato applicato per parecchi anni questo ha dato luogo a sistemi di corruzione

Per tali motivi, non avendo ad oggi indirizzi diversi da parte del Ministro, rispetto all'impianto normativo di questo provvedimento, ho espresso il mio favore in ordine a questo articolo nelle sue varie esplicitazioni.

quali agli annunci non seguivano i fatti promessi, fa un salto di qualità. Oggi siamo arrivati alla politica dell'annuncio cui seguono fatti diametralmente opposti rispetto all'annuncio medesimo. un annuncio molto chiaro già il nome del partito maggiore di Governo: Popolo della Libertà; ora sarà bene integrarlo: Popolo della Libertà,

l'Italia in Europa e nel mondo, a rendere l'Italia un Paese capace di competere nell'arena internazionale. dire questo al seminario di Cernobbio, davanti alla stampa internazionale e ai protagonisti dell'economia globale, perché sapeva che la scelta di limitare la concorrenza è contro il parere dell'Antitrust, contro il parere e l'indicazione precisa dell'Unione europea; sapeva che probabilmente questa norma verrebbe cassata dalla Corte di giustizia europea;

Attenzione: il processo del lavoro è gratuito solo nel senso che l'imposta di bollo sugli atti giudiziari è azzerata, ciò non significa certo che gli avvocati che si occupano di diritto del lavoro non si facciano pagare; non significa certo che le tariffe minime che state reintroducendo non si applichino nelle cause di lavoro. Se è questo ciò che vuol dire, senatore Mugnai, mi sembra che stia prendendo un grosso abbaglio, stia dicendo una cosa non vera. Nelle cause di lavoro gli avvocati si fanno pagare eccome. L'altra obiezione è quella secondo cui,

con partecipazioni agli utili, cioè con forme di retribuzione che, pur riferite a prestazioni di mezzi, sono correlate al risultato della prestazione. Anche questa obiezione del senatore Mugnai non sta in piedi. A questo punto mi chiedo se davvero abbia un senso che con motivazioni così deboli, che non stanno in piedi, voi continuiate a difendere una disposizione che ci fa fare un pesante passo indietro rispetto al resto d'Europa e che, oltre tutto, ci pone in contrasto con precise disposizioni *antitrust* dell'ordinamento europeo e dell'ordinamento nazionale.

che per una professione liberale non ci debba essere tariffe minime imposte per legge, e ancora meno possano esserci tariffe massime imposte per legge, e di cui non Questa è la ragione: non perché c'è l'*Authority*, la quale deve governare se stessa e quindi fa un'autoapologia sull'*how to*, come si usa, e neanche per quello che dice la Comunità europea. Tanto meno capisco il divieto del patto di quota lite, un fenomeno che, oltre a quel che ha detto il professor Ichino, non vedo caratterizzato dalle prerogative negative espresse dal Sottosegretario.

Abbiamo sentito le motivazioni del Governo e del relatore sull'abolizione del patto di quota lite. Io non ritengo di dover dire come la penso in merito, anche perché mi asterrò dal voto, ma una considerazione va fatta, perché qui siamo in sede legislativa. Non bisogna essere magistrati, avvocati e cultori del diritto per capire questo gioco, questa ipocrisia normativa. Si abolisce il patto di quota lite 12.8, alla lettera *c)*, che la maggioranza si appresta a votare, che le parti possono prevedere «un premio in caso di esito positivo della controversia o per il caso di conciliazione».

**Il Senato non approva.**

la reintroduzione delle tariffe minime e registriamo che su questo punto, che già suscitò un dibattito molto esteso sia in Parlamento che nel Paese, non c'è un avvicinamento tra le due posizioni che vengono Cito per tutti il senatore Caruso, che ha ricordato questa mattina gli argomenti a sostegno della tesi della maggioranza nei modi che abbiamo ascoltato, e quelli che sono stati svolti da molti colleghi del nostro Gruppo. gli argomenti che sostengono le rispettive posizioni. C'è un aspetto che riguarda la derogabilità delle tariffe minime su cui ci si potrebbe invece trovare tutti quanti d'accordo: riferisco al fatto che la derogabilità delle tariffe minime aiuterebbe indiscutibilmente l'accesso dei giovani professionisti al mercato dei servizi legali. Su questo non ci sono dubbi. Comprendo la ragione esposta in base alla quale i grandi gruppi, le banche e le compagnie (cioè chi ha un'elevata forza contrattuale), attraverso l'utilizzo della norma che era stata approvata nel 2006, cercano di fare gli affari propri, abbassando fino abbassando fino al limite della sussistenza i compensi per i professionisti. Ma non c'è alcun dubbio che attribuire a questo mercato

Lo so bene che lo vogliono evitare, ma abbiamo ascoltato gli argomenti. Qualcosa la dobbiamo però pur fare, se è vero, come è vero, che la soluzione che voi state proponendo e che

stiamo tornando indietro di alcuni lustri, quando il tariffario forense per la medesima attività prevedeva che, qualora l'attività fosse svolta dal procuratore legale, la tariffa era ridotta della metà. Questo sistema è poi cambiato, perché è sparita la figura del procuratore e si è deciso che, nel momento in cui l'esame di abilitazione consentiva di svolgere determinate attività, vi fosse un tariffario per l'attività dell'avvocato. caso si introduce, invece, un tariffario diverso per l'avvocato giovane. Si stabilisce, infatti, che il compenso giusto è quello previsto per l'avvocato:

dobbiamo difendere determinati principi e prerogative introdotti con la riforma della professione forense, e quindi anche dell'esame, che è avvenuta anni fa. fa. Non possiamo consentire che, se è giusto un tariffario minimo per una determinata attività, possa introdursi, solo perché il soggetto debole, in questo caso l'avvocato giovane, è

eventuali deroghe, ma non introduciamo il principio di deroga ad un principio che è più nobile: quello della giusta retribuzione a parità di prestazione.

che non occorrono fondi spese, ma ha detto che non occorre anticipare fondi spese vive in quanto le spese vive non ci sono; vive non ci sono; ha detto questo secondo verità. Altra è la questione della soccombenza: come in qualunque controversia, quando si soccombe, a meno che non si abbia assoluta sfiducia *a priori* nella magistratura giudicante, ci può essere, in base alla valutazione - peraltro discrezionale

un compenso, una retribuzione *intuitu personae*: praticamente, la retribuzione è più vile, più scadente, più modesta, più limitata perché la prestazione viene fornita da un giovane professionista. Come giustamente ha ricordato il collega Li Gotti, abbiamo fatto un percorso per affermare che, dopo un severo, selettivo e valido percorso di preparazione professionale, una volta superato l'esame professionale, non ci sono né *peones* né distinti: ci sono professionisti; è stato unificato l'albo: ci mancherebbe altro che noi dovessimo differenziare la retribuzione prendendo a misura egli anni di iscrizione all'albo forense.

svilire i giovani professionisti, abbandonarli alla mercé di un mercato vessatorio, che farebbe fare un salto all'indietro al percorso virtuoso che è stato innescato in favore della preparazione professionale e dei diritti, non degli anziani,

il diverso trattamento tariffario che avevano i vecchi procuratori legali rispetto agli avvocati. Per i non addetti ai lavori, è bene chiarire: quindici anni fa, l'accesso alla professione forense era articolato in due fasi: la prima era quella

lavoratori parasubordinati di grandi studi legali. Senatori Li Gotti e Benedetti Valentini, andate a chiedere ai giovani avvocati se preferiscono, ad esempio, avere la possibilità di rivolgersi a una banca per dichiararsi disponibili a fare il recupero dei crediti alla metà della tariffa, oppure se preferiscono andare in un grande studio legale a fare lo stesso lavoro ricevendo un compenso vile dall'avvocato titolare dello studio. Credo che non ci sarebbero dubbi. Altro che dignità! Quello previsto dall'emendamento per aprire il mercato a favore dei giovani, per un tempo limitato, trascorso il quale i giovani diventeranno avvocati come gli altri, probabilmente avendo acquisito una clientela e un'esperienza che consentiranno loro di vivere, sotto il profilo professionale, più tranquillamente.

infatti per nulla meravigliato che l'avvocato Longo, che ha un'alta professionalità, si sia dichiarato favorevole all'introduzione del patto di quota lite. non bisogna credere che tutti coloro che possono essere ammessi al beneficio del gratuito patrocinio, che non è una cosa semplice, lo possano fare. L'introduzione del patto di quota lite va a favorire proprio i meno abbienti

Naturalmente, non ci si deve meravigliare che davanti ai giudici del nostro Paese pendano 5 milioni di controversie civili: civili: se l'avvocato, come diceva il senatore Mugnai, non deve essere pagato per il risultato ma per la prestazione, non ci sarà avvocato

Ecco la ragione per cui è stato ritenuto importante nella precedente legislatura introdurre il patto di quota lite:

è questo che alza il livello di professionalità e può contemporaneamente abbassare il numero di cause civili pendenti davanti ai giudici, il che sarebbe veramente essenziale per quella giustizia rapida che tutti invocano.

...non ho capito per quale motivo essere contrario al patto di quota lite significa avere una bassa professionalità e essere favorevoli significa avere un'alta professionalità. Questa è un'impostazione di principio. L'emendamento

prevedeva il divieto del patto di quota lite, salvo un'eccezione...

un'altra, che è ancorata ad una visione di professionalità alta. Allora io dico che sono per le professioni coerenti. Ecco perché ho smarrimento. Non riesco a capire questi richiami etici alla professionalità alta quando qui vedo scritte due cose diverse. Questa era l'opinione che volevo esprimere per giustificare lo smarrimento che mi ha colto nel sentire le motivazioni a proposito dell'emendamento 12.226.

Presidente, se ho ascoltato bene il parere del relatore, che mi invita al ritiro,

Allora, siccome vi sono gli atti parlamentari a dare anche la lettura dell'interpretazione della volontà del legislatore, se siamo d'intesa che, effettivamente, il mio emendamento è ridondante e superfluo, nel senso che la normativa che noi variamo supera quella di cui io proponevo la espressa abrogazione, se siamo d'accordo in questo senso, io aderisco alla proposta di ritiro dell'emendamento. Dobbiamo, però, essere ben chiari nella interpretazione della volontà del legislatore.

che la maggioranza ha votato precedentemente contro un emendamento, il 12.14, con il quale noi avevamo proposto che fossero nulli gli accordi che coinvolgono l'interesse personale dell'avvocato in modo tale da influire sulla sua indipendenza.

rivolgere una garbata replica alla collega Incostante. Esiste il codice deontologico che regolamenta tutte queste incompatibilità. Non è che possiamo inserire nella legge ciò che è già contenuto in un altro provvedimento vincolante. Capisco l'esigenza politica di sottolineare taluni aspetti aspetti delle proposte non accolte, ma esistono delle realtà che - ahimè - confliggono con queste suggestive formulazioni, delle quali dobbiamo prendere atto.

Signor Presidente, l'ordine del giorno G12.200 investe proprio la questione che è stata al centro del nostro dibattito oggi: cioè se davvero la dignità di un mestiere o di una professione possa essere misurata o difesa da una tariffa minima fissata per quel mestiere o quella professione. Su questo punto l'Autorità *antitrust* si è pronunciata in modo molto chiaro. Cito testualmente: «Il decoro è un concetto di valore etico che può essere utilizzato quale principio generale dell'attività professionale, ma non come parametro economico di determinazione del compenso». del compenso». Questo significa che la dignità, il decoro della professione non possono essere difesi limitando la competizione libera in un mercato ben funzionante. Salvo che questo è un punto che deve essere molto chiaro - quel mercato soffra di distorsioni che ne impediscano il corretto funzionamento.

per l'esistenza di precise distorsioni di quel mercato determinate da asimmetria informativa e/o dalla struttura di monopsonio che quel mercato molto sovente assume, cioè l'esistenza di un unico compratore con una pluralità di venditori di lavoro, cosa che determina uno squilibrio di potere contrattuale tra le parti.

davvero non vedete quanto lede il prestigio dell'avvocatura il fenomeno che è sotto gli occhi di tutti, che tutti conosciamo, di avvocati che lucrano proprio in virtù delle tariffe minime delle vere e proprie rendite che talvolta sono colossali? Mi riferisco alle cause seriali,

Credo che la dignità della professione non fosse certamente favorita dalla percezione di quelle rendite. Viceversa, non vedo niente di indecoroso nel

sotto delle tariffe. Ma che cosa c'è di indecoroso in questo? Ci sono interi stuoli di avvocati, in Italia, che lo fanno molto decorosamente e amati e stimati dai lavoratori che si rivolgono a loro. Vengo ora all'obiezione secondo cui nel processo del lavoro non si pagherebbero fondi spese. Certo, non c'è l'esborso per i bolli sugli atti giudiziari, ma l'onorario dell'avvocato c'è e di ciò abbiamo discusso. In questo settore, i minimi professionali vengono diffusamente trasgrediti, solo che non lo si dice. Allora, poiché il riferimento alla dignità e al decoro è del tutto fuori luogo, vi invito a considerare questo ordine del giorno e preannuncio il voto favorevole su di

riconosco la delicatezza della normativa specifica contenuta in questo articolo: come assicurare, attraverso il sistema delle tariffe di un'attività professionale così importante, la qualità del servizio prestato, una dignitosa remunerazione dell'attività forense, un accesso al mercato che assicuri il ricambio della professione. È materia delicata, che francamente non si può affrontare con la semplificazione che spesso c'è in questo dibattito. Anche i confronti che si fanno con gli altri Paesi richiedono la consapevolezza che, oggettivamente, la situazione italiana è diversa, in quanto c'è una particolare aspetto è quello della numerosità.

La seconda pressione competitiva è altrettanto importante e non ne ho sentito assolutamente parlare. Cari colleghi, in Italia sta succedendo un fenomeno che si fa finta di non vedere: il mercato dell'avvocatura non è più un mercato nazionale ma globalizzato il nostro Paese - guardatevi i dati dell'ISTAT- dimostra per il settore dei servizi professionali uno sbilancio commerciale di dimensioni colossali, tra 5 e 6 miliardi di euro, il studi professionali esteri entrano in Italia e competono sul mercato italiano. E qui non potete mettere le barriere! È giusta e legittima la preoccupazione della professione:

Non è la legge che crea la difficoltà, non sono le regole ma è il mercato che è cambiato. E dobbiamo fare delle buone e sagge regole, idonee ad affrontare lo svolgimento della professione in un mercato completamente cambiato.

non si può più immaginare un sistema di tariffe innovative. Ricordo che ci sono professioni, che assicurano redditi elevati, in cui il sistema delle tariffe minime non esiste e gli ordini hanno accettato che non esista più il sistema delle tariffe minime.

nella classifica della regolamentazione della professione: prima la Turchia, poi l'Italia. Dopo questa legge saremo primi, naturalmente: ma vi sembra che sia questo il modo di affrontare i problemi? Gli avvocati non staranno meglio e soprattutto, in compenso, peggiorerà la funzionalità della giustizia. Una cosa è certa: il professionista non potrà competere sulle tariffe; non potrà competere sulla qualità, perché non può fare la pubblicità comparativa, non può far conoscere la qualità dei propri servizi; non può competere sull'organizzazione, perché impedite di fare le società professionali. Su cosa sarà ridotto a competere? Ci sono studi precisi della Banca d'Italia che lo dimostrano: con questo sistema tariffario tentando di innalzare la litigiosità, di prolungare i processi, di moltiplicare gli atti. Ma a voi sembra - lo dico al Sottosegretario, che dice che queste norme servono per la dignità e la trasparenza della professione professione - che professionisti ridotti ed obbligati a fare questo abbiano più dignità, possano tutelare la dignità professionale, migliorare l'efficienza del sistema giustizia, possano dare un miglior servizio al cittadino? È esattamente il contrario. Parlate di riforma della giustizia e attraverso questo arretramento di vent'anni ponete i presupposti perché ancora una volta il servizio della giustizia sia lungo, oneroso per il cittadino, inefficiente per il Paese. E dunque la competitività generale del Paese, come dimostrano tutti gli studi economici, andrà ancora indietro: un buon risultato!

a pagina 42 del testo al comma 6 è inserita anche la clausola «con esclusione della natura subordinata del rapporto» che va eliminata. È un errore materiale materiale evidente, che potrebbe determinare un contrasto con il successivo comma 7 della norma che si propone. Chiedo innanzitutto la modifica del testo. Vorrei sapere se ci sono problemi o se lo posso illustrare.

Presidente, con l'emendamento vogliamo mettere in luce che vi sono gravi difficoltà nell'esercizio della professione di avvocato da parte dei giovani avvocati. Noi non intendiamo avallare un sistema che prevede una forma di sfruttamento delle prestazioni professionali dei giovani avvocati o di avvocato in generale nei confronti di altri studi professionali o di altri avvocati.

con un riconoscimento, quindi, attraverso un tipo di contratto che, in questo caso, può non essere di lavoro subordinato, ma che consenta di avere delle tutele. In caso contrario, giovani avvocati o avvocati meno giovani si trovano nella situazione di non poter contare non poter contare su un introito mensile, di non poter regolare il loro lavoro e la loro vita. Questo influisce negativamente sulla dignità della funzione stessa che viene esercitata. A questo punto aggiungiamo anche la possibilità che la collaborazione continuativa tra avvocati, ovvero tra avvocato e associazioni o società di avvocati anche multidisciplinare, possa dar luogo a rapporto di lavoro subordinato. Non si tratta di una clausola di obbligatorietà, ma di una facoltatività che regolarizza, ancora una volta, un rapporto che esiste tra il professionista e una società di cui entra a far parte, cosa che è riconosciuta negli altri ordinamenti regolarmente. Non si incide assolutamente sull'autonomia dell'esercizio della professione, ma si vuole solo regolarizzare una condizione che non è accettabile. È stato organizzato su questo punto addirittura un convegno di avvocati

né, a maggior ragione, da un lavoro dipendente, che da loro viene sollecitato ed accettato senza alcuna limitazione di autonomia, ha messo in luce le gravissime condizioni in cui versa buona parte dell'avvocatura italiana e, soprattutto, le fasce giovanili dell'avvocatura italiana. Siccome vogliamo risolvere questi problemi, non bloccare il futuro dei giovani ed anzi consentire loro di poter avere un futuro migliore nel loro interesse e nell'interesse della società italiana, riteniamo che questo emendamento debba essere approvato.

diversa formulazione, dall'articolo 4 del decreto legislativo n. 96 del 2001, che si occupa specificamente delle società di professionisti. Sono dell'opinione che le due norme debbano viaggiare indipendentemente. Vi sarà poi un momento in cui, è auspicabile che sia, verrà formato un testo unico che regolamenti la professione, ma fintanto che ciò non avvenga sono dell'opinione che è bene che le due norme rimangano distinte tra loro.

non dà mai luogo a rapporto di lavoro subordinato». Oggi questa è la norma che regola la materia; quindi questo comma non introduce una novità. Tuttavia, il ribadire questa norma contrasta con un orientamento molto preciso della Corte costituzionale, che stabilisce che il legislatore ordinario non può *facere* *de* *albo* *nigrum*, ovvero stabilire che è autonomo ciò che è in realtà subordinato. La Corte costituzionale stessa avverte che ci possono essere molti buoni motivi, in situazioni particolari, per modificare la disciplina del rapporto in questione

al regime di assicurazione della cassa avvocati e non al regime dell'assicurazione generale INPS; oppure dettare norme particolari in materia di licenziamento per non assoggettare il rapporto allo Statuto dei lavoratori. Tutto ciò è perfettamente legittimo, dice la Corte costituzionale, ma quello che non si può fare è dire che è autonomo ciò che in realtà è subordinato. allora perché dobbiamo commettere qui un errore tecnico quando la Corte ci ha indicato in modo molto preciso e limpido

che si determini un vero e proprio rapporto di dipendenza; ci sono praticanti che sono molto più subordinati e molto più dipendenti di quanto non sia un normale lavoratore subordinato.

che è evidentemente sbagliato e incostituzionale, e sostituiamolo con una normativa adatta alla specialità del rapporto.

Facciamo un'operazione di questo genere anche per quelle posizioni tipiche del lavoro forense che hanno tutti i caratteri della subordinazione e che per certi aspetti meritano anche una qualche tutela tipica del lavoro subordinato, ma che è tuttavia giusto esentare dalla disciplina generale del lavoro subordinato. Credo che in proposito non ci siano problemi di destra e sinistra, di maggioranza e opposizione, e neanche problemi di favore nei confronti di un'istanza della professione forense rispetto a interessi sottolineati dall'Antitrust o da altri enti esponenziali. Si tratta solo di una questione di correttezza giuridica e di buona tecnica legislativa, la quale ci evita di andare contro un orientamento costituzionale che è ben conosciuto e ribadito in numerose sentenze. Per queste ragioni, propongo di concordemente il comma 4 e magari, con l'accordo del relatore, individuare gli emendamenti integrativi che possono adeguatamente sostituirlo.

così come proposta dal relatore e dal Governo in questo momento, stabilisce che gli avvocati possono farsi sostituire da altro avvocato con incarico, anche verbale, e la delega scritta è riservata soltanto ai praticanti abilitati. Riteniamo che questa norma debba essere collegata al successivo comma 3, nel senso che, quando si tratta di sostituzioni, rimane comunque la responsabilità personale dell'avvocato cosiddetto delegante nei confronti dei clienti. Riteniamo che la chiarezza, una maggiore trasparenza e il senso di responsabilità debbano imporre una delega scritta. Abbiamo inserito tali previsioni nel nostro emendamento principale,

stabili. In proposito, l'emendamento 13.210 prevede appunto la possibilità per l'avvocato di nominare sostituti stabili,

che chi subisce un danno da determinate vicende sia soltanto il cliente, senza possibilità di riconoscere immediatamente, in maniera chiara e trasparente una responsabilità per l'avvocato delegante. In questo senso, quindi, vanno i due emendamenti

dalla seconda parte del comma 6, che prevede che «Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro della giustizia di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze ed il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentita la Cassa nazionale di previdenza ed assistenza

gli Uffici mi informano che non è una questione di forma, ma di sostanza. Credo tuttavia che sia bene, poiché non c'è la motivazione, che la Commissione bilancio o il suo Presidente si esprima si esprima in particolare per quanto riguarda l'eventuale modifica del comma 6, così come lei l'ha proposta per

Chiedo pertanto alla Commissione bilancio, al Presidente o al Vice Presidente, di esprimersi in questo senso; altrimenti evidentemente sarò costretta ad accantonare

prevede delle modifiche alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale in materia di elenchi e tabelle dei difensori d'ufficio. Noi parliamo quindi di difesa d'ufficio; è evidente che trattandosi di una materia così delicata, l'intervento da parte del Ministro della giustizia, sollecitato

aggiornamento di albi, elenchi e registri. In questo caso, si richiede infatti che l'albo, gli elenchi e i registri siano a disposizione del pubblico e siano pubblicati nel sito Internet dell'ordine, fatto che ogni comunicazione di variazione sia data agli uffici giudiziari interessati. Questa è la ragione dell'emendamento: l'impalcatura della legge, ma intendiamo dare al Ministro un potere di intervento complessivo di carattere generale nel settore, mettendo contemporaneamente gli uffici giudiziari

dall'esercizio professionale per qualsiasi causa, che deve essere indicata, ed inoltre degli avvocati cancellati per mancanza dell'esercizio continuativo della professione, nonché l'elenco degli avvocati che hanno subito provvedimento disciplinare non più impugnabile, comportante la radiazione». In buona sostanza, questo aspetto, che mi pare particolarmente significativo e che afferisce ad un'area circoscritta di avvocati

se ho capito bene, il relatore stima utile implementare la disposizione come ora prevista con

Accetta la riformulazione

è opinione diffusa che meriti un approfondimento, poiché il sistema attuale non garantisce un'effettività di difesa, crea un sistema terziario di lavoro

se non ricordo male, non tutti gli avvocati potranno essere nominati difensori d'ufficio come avviene oggi, ma solo quelli specialisti, cioè quelli che si iscriveranno nell'apposito elenco dei penalisti. Questa scelta in linea generale può essere condivisibile, perché se facciamo una riforma che tende a stimolare, favorire e promuovere la specializzazione tra avvocati è giusto che i processi penali siano svolti innanzitutto da chi è specialista, quindi da chi è penalista. Sennonché, per i giovani avvocati l'acquisizione di questo titolo specialistico richiede molto tempo,

questo articolo, così come ci viene proposto, sarebbe preclusa ai giovani avvocati la possibilità di fare i difensori di ufficio. Oggi, per moltissimi giovani avvocati, l'attività di difensore di ufficio è diventata quasi l'attività prevalente, perché è una di quelle attività che si svolge

non superi i tre anni - sia possibile nominare i giovani avvocati difensori di ufficio, come avviene oggi per tutti i reati. oggi per tutti i reati. Oggi, un giovane avvocato, anche se non è penalista, in teoria, se chiede di essere iscritto in un elenco, può chiedere e ottenere di essere nominato difensore di ufficio anche per un reato di omicidio, per un reato di mafia, per un reato gravissimo.

Quando c'erano le preture, signora Presidente (periodo che io ricordo perché all'epoca ero un giovane avvocato), si potevano patrocinare davanti alle preture, da praticante, non solo le cause penali: il praticante

ai giovani avvocati anche di fare i difensori di ufficio. È troppo! Ripensate almeno a questo, perché tale emendamento non cambia la sostanza del provvedimento. Esso assicura la specializzazione, va nella direzione auspicata ma, almeno, consente, per i reati

si debba ripristinare lo *status quo*, nel senso di consentire a tutti gli avvocati di accedere all'incarico di difensore di ufficio. Però, prendendo atto che si vuole riservare questa attività agli specializzandi, bisogna porre un termine.

dopo di che compirà i cinque anni per fare l'esame e diventare specialista: come minimo occorrono sei anni. Di qui la ragione dell'indicazione del termine di sei anni.

del collega Legnini, il quale ha ricordato la figura del pretore e del praticante procuratore che poteva esercitare davanti al pretore. Il pretore, signora Presidente, è una figura rimpianta. Io che votai contro quella riforma ricordo con quanta tenacia cercammo di salvare quella figura, che

importanza, francamente mi induce perplessità. Le devo questa risposta, senatore Legnini, per il rispetto che debbo alla puntualità con la quale lei sempre argomenta le sue proposizioni; però mi pare che proprio la situazione particolare che si viene a creare nel giudizio davanti al giudice di pace impone la piena consapevolezza che vi siano capacità, responsabilità e consapevolezze da una parte e dall'altra dei banchi. Per questa ragione, ahimè, sono costretto a confermare il mio parere contrario.

indubbiamente un punto di grande rilievo. Tuttavia, manifesto una perplessità e il mio voto è condizionato dal perdurare di questo mio dubbio.

Ma non c'è scritto «anche». Si dice che per quella fascia di reati i difensori d'ufficio possono essere esclusivamente quelli iscritti all'albo da non più di sei anni, il che significa che quelli che sono iscritti da sette anni non possono assumere quelle difese.

Non siamo certo noi a fare ostruzione, stiamo solo affrontando un problema concreto. Il collega Legnini, contro le cui tesi ho parlato poco fa, in questo caso prospetta una cosa che - come diceva il senatore Li Gotti - ha una sua concretezza. La vera domanda domanda è: vogliamo trovare una forma che, almeno nel settore della difesa d'ufficio, agevoli o dia una corsia preferenziale ai giovani professionisti? Diciamolo fuori dai denti: la domanda sarebbe questa.

avvocati iscritti in quell'anno, anche perché - come ricordavano i colleghi - lei sta implicitamente inibendo la possibilità di essere nominati d'ufficio a coloro che hanno un'anzianità di iscrizione superiore ai sei anni.

ad accogliere il suggerimento del senatore Li Gotti. Non intendevo dire che solo i giovani avvocati fanno quel mestiere, ma che anche i giovani avvocati possono farlo, perché non si capisce la ragione per cui dobbiamo vietarglielo.

che nell'economia di questo provvedimento ha un suo rilievo. Questo disegno di legge è in gran parte mirato a scoraggiare i giovani dal fare l'avvocato: neanche su queste cose riusciamo ad interloquire, non va bene. Faccio notare al relatore, senatore Valentino, che la sua tesi è molto singolare: di fronte ad un giudice ad un giudice onorario, che tratta delle questioni minime, quotidiane, despecializzato (in genere è un funzionario dello Stato o un avvocato in pensione che, come sappiamo tutti, va a fare il giudice di pace), secondo lui dovrebbe esserci il principe del foro.

Nessuno: i grandi avvocati ci mandano i praticanti, come sappiamo tutti, e poi percepiscono l'onorario al massimo livello.

La domanda che pongo agli esperti - perché è talmente da esperti questa materia che si fa fatica a starci dietro - è questa: nel momento in cui andiamo ad introdurre la tariffa minima, cosa succede dal punto di vista della copertura per il patrocinio gratuito? Noi diciamo che si introduce una tariffa minima. Il patrocinio gratuito sta esplodendo, lo Stato non ha i soldi per pagarlo. Giustamente viene detto: almeno favoriamo i giovani! Prima abbiamo detto però di non favorire i giovani per legge. Probabilmente, se lasciamo fare al mercato è meglio, ma questa è una mia banale considerazione. Però, visto che avremo modo di tornarci, chiedo ai colleghi più esperti se ci possono dare qualche lume su una questione di di una qualche rilevanza in tema di copertura di tutto il provvedimento.

Presidente, mantengo le mie perplessità. Innanzitutto i procedimenti sono quelli di competenza del giudice di pace e del tribunale. L'emendamento anche questi procedimenti propone, anche se poi la pena edittale non può essere superiore a tre anni. Ma il fatto che sia prevista la competenza del tribunale, già questo presuppone una oggettiva, intrinseca gravità dei fatti dei quali si discute. Noi ci stiamo preoccupando di garantire la massima professionalità a coloro che sono posti davanti alla giustizia. Capisco perfettamente che bisogna trovare una sintesi fra tante esigenze e che bisogna guardare con grande attenzione alle ragioni dei giovani avvocati che si avviano alla professione. Però mi pare che l'esigenza di tutelare rigorosamente la competenza prevalga su tutto. E il disegno di legge, così com'è formulato, quell'esigenza tutela. E di quel disegno di legge si è discusso nel corso degli incontri che abbiamo avuto con tutti i rappresentanti istituzionali dell'avvocatura, le associazioni di categoria e in particolare la camera penale. Quindi, pur rendendomi conto dell'importanza del tema che viene sollevato dal senatore Legnini, debbo confermare il mio parere contrario. PRESIDENTE. E il Governo?

vorrei proporre l'accantonamento di questo emendamento perché il senatore Valentino possa riflettere anche sugli argomenti dei senatori Benedetti Valentini, Longo e di altri colleghi che credo per larga

Presidente, non mi unirò alla maggioranza per far accantonare l'emendamento 15.206, però in effetti il comma 3 dell'articolo 15 recita: «Le disposizioni di cui al comma 2» - che abbiamo già adottato - «si applicano a decorrere dal quarto anno successivo all'entrata in vigore della presente legge».

- sapete che la legge professionale forense attuale prevede come requisito per l'iscrizione all'albo la cittadinanza italiana. Ovviamente, a seguito anche dell'applicazione dell'ordinamento comunitario, il requisito è stato interpretato in senso estensivo ammettendo l'iscrizione all'albo anche di cittadini di Stati membri dell'Unione europea. Ma si è sempre pacificamente riconosciuto che un cittadino straniero non poteva essere iscritto all'albo degli avvocati. Questo è congruente con un modello di avvocato che abbiamo scelto consapevolmente, cioè con un modello di avvocato che esercita delle funzioni pubblicistiche. Abbiamo prima detto che l'avvocato ha una funzione sociale e una funzione pubblica. Abbiamo scartato un modello che che vede nell'avvocato un mero prestatore di servizi legali che opera in un mercato aperto alle leggi della concorrenza e abbiamo scelto un modello prefigurato dalla Carta costituzionale di un avvocato che esercita una funzione sociale e che, dunque, ha un rilievo pubblicistico. Ecco perché noi chiediamo che venga inserito espressamente fra i requisiti per l'iscrizione all'albo il requisito della cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell'Unione europea. Ci appare un requisito scontato ma che giustamente deve essere espresso nella nuove legge sull'ordinamento forense. Chiudo dicendo che il maestro di tutti noi sull'ordinamento forense che ha scritto un manuale sul tema, dice che la cittadinanza italiana è il requisito richiesto prima di ogni altro per l'iscrizione all'albo degli avvocati. dice che nessuna discussione sembra prospettarsi al riguardo. È un concetto scontato e banale, ma che nell'ordinamento forense nuovo che stiamo scrivendo in questi giorni dobbiamo assolutamente inserire.

eccentrica della quale si stenta a capire la ragione. Mi riferisco all'inserimento di una norma che fa divieto ai professori ordinari in materie giuridiche, ai magistrati (a meno che fosse rivolta ai magistrati e trascini con sé altre categorie) e persino agli avvocati dello Stato che abbiano svolto le funzioni per almeno cinque anni

La norma è ancora più strana perché, come loro sanno, professori e magistrati sono chiamati a comporre le commissioni di esame per l'abilitazione alla professione forense.

qualora decida di cessare l'attività, peraltro pubblica (pensiamo agli avvocati dello Stato che fanno a pieno titolo gli avvocati e quindi rappresentano in udienza lo Stato in vicende molto spesso complesse, per non parlare dei magistrati). Com'è possibile introdurre tale norma addirittura in una prima fase? Ne

emendamento il ripristino di una situazione credo ispirata alla ragionevolezza, al buon senso e anche al rispetto per il lavoro che alcune figure individuate svolgono nella loro attività.

la cancellazione d'ufficio dagli albi, elenchi e registri quando viene accertata la mancanza del requisito dell'esercizio continuativo della professione ai sensi dell'articolo 20.

riteniamo che tale requisito della continuità della professione non possa costituire requisito dirimente ai fini della permanenza nell'albo degli avvocati. Abbiamo già discusso in riferimento ai primi articoli di questa legge su questo punto e abbiamo tra l'altro osservato che il requisito della continuità è incompatibile con un divieto di discriminazione indiretta ai danni delle lavoratrici, in questo caso delle avvocatesse, perché è noto che nell'attività lavorativa delle donne la discontinuità è statisticamente maggiore rispetto agli uomini. Sulla base di questa osservazione statistica, la Corte di giustizia ha vietato tutte le clausole di regolamenti, contratti collettivi o leggi che condizionino alla continuità, o ad un certo tasso di continuità, Questo significa che noi non possiamo introdurre un criterio di continuità senza determinare un danno, un pregiudizio, per la parte parte femminile della platea a cui la norma si riferisce: in questo caso, la platea degli avvocati. Questo è il motivo per cui proponiamo la soppressione di questa disposizione naturalmente torneremo su questo punto quando arriveremo all'articolo 20.

nella discussione precedente (che ha portato all'accoglimento da parte della maggioranza del suggerimento contenuto nell'emendamento), l'omesso riferimento al procuratore della Repubblica presso il tribunale e al procuratore generale presso la corte d'appello è il risultato

tratti di un errore omissivo, perché mi trovo davanti a una maggioranza che non si stanca di ripetere che questo Governo e questa maggioranza combattono la mafia più di qualsiasi altro Governo del passato.

nascosto, ma che va risolto. si dimentica che i professori di ruolo delle università dello Stato dei settori scientifico-disciplinari di area giuridica possono non essere, e ciò spesso avviene, non laureati in giurisprudenza.

perché fa riferimento ai requisiti del comma 1, lettere *b)*, *c)*, *d), e)* ed *f)* e non all'articolo 2, che è stato votato questa mattina e che fa presente che devono essere laureati in giurisprudenza.

è fondamentale, perché riguarda i criteri di iscrizione e di cancellazione dall'albo, e quindi vi è un'articolazione abbastanza specifica però dei punti critici. Dobbiamo riconoscere che questo è stato uno degli argomenti che più ci ha impegnato in Commissione, perché le perplessità e i punti di criticità sicuramente permangono. Sono d'accordo con il senatore Maritati e quindi anche con i proponenti degli emendamenti circa il fatto che si debba prevedere una specificazione delle cause preclusive all'iscrizione all'albo per reati gravissimi, per i quali, nella gran parte dei casi, è prevista l'interdizione perpetua dai pubblici uffici,

ma si potrebbe assumere il ruolo di difensore d'ufficio, che obiettivamente è un pubblico ufficio in quel momento, pur essendo interdetto permanentemente. Si creerebbe in questo modo una situazione di grave contrasto strutturale: è impensabile che l'interdetto in maniera perpetua possa assolvere alla funzione di difensore d'ufficio, svolgendo una funzione che viene così prevista e disciplinata da questo impianto legislativo. Sulla struttura generale dell'articolo 16, quindi, indubbiamente vi è una condivisione tranne questi interventi specifici, che devono coordinare alcune previsioni con altre relative ad altri settori del nostro ordinamento: l'armonia è sempre necessaria quando si interviene nel riconoscere dei diritti che scaturiscono da una iscrizione e le conseguenze che scaturiscono da una cancellazione. Stiamo affrontando il tema dei diritti, ma dobbiamo armonizzarli con il nostro sistema, che è fatto anche di altre regole e di altre norme,

priva di effetti rispetto alla previsione più vasta che avevamo avanzato, ma non avrei difficoltà a modificare il mio emendamento in tale direzione.

a conclusione della seduta antimeridiana di domani si riunirà la Conferenza dei Capigruppo per organizzare i tempi del seguito dell'esame del disegno di legge di riforma della professione forense a partire dalla settimana prossima.